La seduta è aperta *(ore 11).* Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 ottobre 2017. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, occorre approvare il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 ottobre.

PLI))*. Signor Presidente, i senatori del nostro Gruppo, ovviamente con il massimo rispetto per chi si esprimerà diversamente, pensano che questo che questo sia stato uno dei provvedimenti più sconclusionati, più contraddittori, peggio pensati e peggio scritti che siano giunti all'attenzione dell'Assemblea.

Probabilmente, in casi simili - come ripetutamente ci ha ricordato la collega Mussini - la legislazione italiana viene brillantemente in soccorso di atteggiamenti del genere, perché stabilisce la distinzione tra le segnalazioni e le denunce. Francamente è un confine molto ipocrita, del tutto fuori dal nostro ordinamento costituzionale, del tutto estraneo allo Stato di diritto.

il pentitismo. Tuttavia, nonostante la retorica e l'ipocrisia di tanti sacerdoti dell'antimafia, la memoria storica del Paese deve saper essere attenta. Il pentitismo (Governo Spadolini) nacque per far fronte al terrorismo, al rapimento del ragazzo Peci, fratello del più noto brigatista

su «Il Foglio», a un certo punto diceva che la delazione può essere una tragica necessità in una Repubblica anche ben ordinata, per esempio in materia di terrorismo. Eravamo al principio degli anni Ottanta quando fu varato il primo esempio di legislazione premiale. legislazione premiale. Su quello che ha significato la legislazione premiale il Parlamento ha rifiutato di indagare: non c'è mai stato all'ordine del giorno di nessuna Commissione antimafia, nelle ultime sette, otto legislature, un'inchiesta sul pentitismo, sui suoi frutti tossici e sui suoi frutti ben riusciti (ci possono essere e ci sono certamente anche quelli).

la delazione, le attribuisce un valore assoluto, non relativo, e si riempie le guance della più insulsa retorica contro contro la corruzione, ovviamente la corruzione percepita, all'indomani di un fallimento legislativo terribile,

un uno strumento legislativo per espellere dal Parlamento il capo dell'opposizione. Nella discussione di ieri, ad un certo punto, erano in gioco diritti costituzionali fondamentali: quello al giusto processo e quello alla difesa. Il senatore Palma ha provato timidamente a ricordare al relatore come questi principi debbano essere di rango superiore alla segnalazione, se non vogliamo dire alla delazione, ovvero al regime di particolarismo giuridico in cui andiamo a collocare il segnalante nel luogo di lavoro ed anche al di tutto questo è avvenuto nell'indifferenza, forse addirittura nella insofferenza del relatore e da questo punto di vista, signor Presidente, al di là del merito del provvedimento contro il quale voteremo,

in Commissione giustizia sono stati elegantemente bypassati attraverso la formula - per carità, più che legittima - del comitato dei pareri. Detto questo, non si è mai avuta l'impressione, in quest'Aula, che né da parte del relatore, né da parte del Governo si sia cercato di ovviare a questa caratteristica. Assistiamo quindi, in un ultimo frammento di retorica contro la corruzione (quella percepita) ad un altro piccolo spicchio di legislazione premiale, mentre ci siamo preclusi

si fa molto di peggio: si introducono come elementi di vita quotidiana il ricatto e la ricattabilità e si rende odiosa la convivenza fra cittadini; e tutto questo senza chiarire nulla degli aspetti strettamente giuridici (da quando fino a quando, che cosa significa questo, che cosa significa quest'altro). Abbiamo provato a chiedere, in questi giorni di dibattito, un minimo di chiarimento e di confronto, e ringrazio in particolare il senatore Malan, che è stato attentissimo e che con i suoi emendamenti ha richiamato la nostra distratta attenzione su molti profili del provvedimento, ma questo è un provvedimento che disonora quest'Assemblea e disonora il lavoro parlamentare. Questa retorica dell'anticorruzione fa parte del pessimo repertorio del moralismo di massa. Nella storia dei Parlamenti c'è un avversario insidioso che va in piazza e si insinua nel senso comune: si tratta del moralismo, quello che ha creato questa odiosa figura del segnalante, del segnalante ricattante

Il denunciante può essere infatti visto come una sorta di traditore, di spia e di certo chi segnala è guardato con diffidenza dalla dirigenza e dai colleghi.

ricondurre tutta la nostra società su binari di perfetta legalità, da conservare a tutti i livelli, all'interno sia di strutture pubbliche che di strutture private.

La qualità della legislazione è fondamentale ed è stato rilevato più volte che la normazione così puntuale, borbonica, piena di incisi e di virgole

all'infamia e alla diffamazione che si può avere in un periodo antecedente, cioè quando viene denunciato il fatto; intendo dire che quando si avvia qualsiasi tipo di procedimento tutti sono sui banchi

e poi, a fronte di questo tipo di interesse, vi è l'esito a volte incerto di una procedura così come viene attivata. Bisogna quindi capire se questa legge ha la capacità di dare equilibrio a tutto ciò

ma sarei tentato di dire che la delazione sia di per sé una manifestazione di scarsa eticità. Ho già ricordato in discussione generale che nel nostro ordinamento ci sono già la legge Severino, due decreti legislativi del 2001 e la normativa che ha istituito l'Autorità anticorruzione a tutelare il pubblico dipendente che segnala i casi di corruzione o altri illeciti sul posto di lavoro: sia nel testo unico sul pubblico impiego sia nel diritto del lavoro si stabilisce che i dipendenti che denunciano reati non possono essere mobbizzati, sanzionati, licenziati, e, se ciò avviene, chi lo fa o commette un reato a sua volta o commette illeciti disciplinari. già leggi adeguate per tutelare il civismo positivo e per punire i reati o gli abusi, nel settore pubblico come in quello privato. Dobbiamo allora chiederci se la legge che vi accingete ad approvare sia veramente necessaria o invece sia l'effetto di una precisa ideologia che nasce dalla cultura del sospetto Il testo, inoltre, contiene evidenti criticità, a partire dalla premialità rispetto a comportamenti che, ove non scorretti, meritano certo una protezione, ma la legge dovrebbe almeno specificare meglio la condotta di abuso oggetto di segnalazione, e delineare in modo più netto il rispetto della presunzione di non colpevolezza. Si esclude l'applicabilità della nuova disciplina alle segnalazioni che configurano il reato di calunnia o diffamazione, ma anche questo è già previsto nella cosiddetta legge Severino. Si vieta di rivelare l'identità dell'autore della segnalazione in assenza del consenso del segnalante e si prevede la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima nei casi in cui essa sia adeguatamente documentata. Ma cosa significa «adeguatamente documentata»? Questa legislatura passerà ormai alla storia come quella che ha introdotto nel nostro ordinamento le fattispecie di reato più vaghe e quindi più pericolose e illiberali, come il traffico di influenze, e io vi invito a considerare quanto possa essere devastante l'introduzione di questo meccanismo di delazione attraverso segnalazioni segnalazioni anonime negli uffici pubblici e nelle aziende private, che prima di tutto comporterà un rallentamento dell'attività amministrativa, in quanto sarà purtroppo inevitabile che vengano aperti anche procedimenti basati più sull'odio e sulla smania di carriera, che sulla sostanza. è inoltre introdotto in questa legge il principio dell'obbligatorietà della denuncia anche nei confronti dei privati cittadini. Ma il nostro ordinamento non prevede che i privati siano obbligati a denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza, tranne nel caso in cui si tratti di reati contro la personalità dello Stato. Questo diritto-dovere non è contemplato, e quando si arriverà all'applicazione concreta di questa normativa si porrà sicuramente il problema della sua incostituzionalità. Si tratta, poi, di norme tutte sbilanciate a favore del denunciante, mentre c'è poco o nulla a garanzia del denunciato. Peraltro, se denunciare è un dovere, perché chi lo fa deve essere premiato?

il giudice ha già in mano tutti gli strumenti per decidere se una denuncia è stata fatta per odio o per invidia, e non per il bene dello Stato o dell'azienda. Dobbiamo chiederci: qual è il confine? Cosa significa che il denunciante ritiene «altamente probabile» che la condotta illecita o l'abuso si sia verificato? In questo modo si sancisce surrettiziamente l'inversione dell'onere della prova, un'aberrazione che in Italia è esistita finora solo nella giustizia sportiva. E pensare che il testo è stato anche migliorato rispetto a quello originario. Ma il meccanismo innescato finirà per non produrre quasi mai effetti negativi sul denunciante, che resterà coperto e al sicuro in tutti i casi in cui non abbia agito con colpa grave, ma, come ho già detto, non è certo semplice specificare cosa sia colpa grave e cosa no. Gli effetti invece saranno pesantissimi sul denunciato, che, per un periodo di tempo indeterminato, si vedrà compromessa la carriera, oltre a finire nel tritacarne della gogna mediatica. La nostra è una Costituzione formale garantista, che tutela la libertà e la dignità delle persone, ma questa parte è stata da tempo soppiantata dalla Costituzione materiale invalsa, visto che la dignità delle persone viene troppo spesso calpestata, ad esempio con la pubblicazione di intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con profili giudiziari; intercettazioni acquisite dallo Stato con i soldi pubblici e utilizzate per distruggere la dignità non solo di persone solo indagate, ma anche di chi non è neppure sospettato di aver commesso reati. Concludo. La *ratio* di questa legge, ossia prevenire i reati e contrastare la corruzione, non può che essere condivisibile, e anche quella di tutelare chi ha il coraggio di denunciare gli abusi, ma il suo contenuto non solo va a peggiorare norme già esistenti, ma rischia anche di scardinare il principio di convivenza sociale e civile, che è uno dei cardini di uno Stato democratico e liberale. Non a caso, in quest'Aula qualcuno ha fatto riferimento a dittature del secolo scorso, che fondavano il loro potere anche sulla delazione. Ma i nostri Costituenti vollero l'Italia come una Repubblica fondata sul lavoro, non certo sulla delazione nei posti di lavoro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mafie e corruzione sono un'emergenza nazionale. Personalmente, io e molti altri senatori in quest'Aula l'abbiamo ripetuto fino alla nausea: ma non basta, evidentemente. Proseguiremo a dirlo e a diffondere il messaggio di Papa Francesco, che ha detto reiteratamente che chi vive di corruzione mangia un pane sporco. Proprio qualche giorno fa Transparency International ha pubblicato il suo rapporto annuale e l'Italia si colloca in posizione imbarazzante per livello di corruzione in Europa. Peggio di noi fanno solo Bulgaria e Grecia. A parole, tendenzialmente, siamo d'accordo tutti. Però, quando, si viene agli strumenti per combattere la corruzione cominciano i distinguo, le cineserie, i barocchismi, in cui gli avvocati sono maestri e le destre diffidenti. Invece, noi dobbiamo essere chiari e determinati nella ricerca e nella pratica degli strumenti per la lotta alla vendita delle funzioni pubbliche, alle clientele, agli abusi e ai favoritismi che minano alla radice il vivere civile e il capitale sociale, che è fatto delle fiducia dei cittadini in se stessi e nelle loro istituzioni. Giovedì, signor Presidente, è stato presentato in sala Zuccari il libro di Andrea Franzoso. Chi era costui? Anzi: chi è? È un *whistleblower*, una persona che per dovere d'ufficio doveva vedere le magagne, le ruberie e la corruzione e non ha girato la testa. Ha preso visione di carte, ha fatto i controlli che doveva fare e ha visto la corruzione in faccia. Ha segnalato a chi di dovere, ma Ha segnalato a chi di dovere, ma quel qualcuno ha girato la faccia dall'altra parte; anzi, lo ha sollecitato a lasciar perdere. Allora lui ha denunciato. ha pagato lui per primo. È ben vero che la persona che lui aveva segnalato quale autore di illeciti è stata condannata. Ma la ritorsione non l'ha risparmiato e lui si ritrova senza lavoro, pur la corruzione, come dicono i penalisti, è un reato a concorso necessario, vale a dire non si può fare da soli. Ci vuole un accordo corruttivo, un corruttore che dà o promette e un corrotto che si fa dare o promettere. I corrotti hanno un patto e il loro interesse è a non denunziarsi a vicenda. Per questo ci vuole un terzo, un orecchio e un occhio neutrale che denunzi se scopre qualcosa, come, per esempio, una cresta su un rimborso spese, un appalto dato senza gara, un collaudo fatto male. Con questo disegno di legge noi vogliamo migliorare la disposizione già introdotta con la legge Severino, rafforzare la tutela dei segnalanti, evitare che le ritorsioni restino impunite, evitare che il *mobbing* e l'isolamento sociale che il denunziante subisce rovinino la sua persona e la sua famiglia. Il segnalante dovrebbe essere, non solo tutelato, ma premiato come si fa negli Stati Uniti. Il percorso dei rimedi contro le ritorsioni deve essere più spedito e sicuro. L'impianto legislativo deve essere un monito per i corrotti, non un percorso a ostacoli per chi segnala. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge e diciamo a tutti gli Andrea Franzoso d'Italia di andare avanti!Lo diciamo al ricercatore di diritto tributario che di recente ha denunziato il verminaio dei concorsi universitari nella sua materia; e lo diciamo a tutti i dipendenti degli enti locali che assistono sconvolti alle ruberie in parecchi uffici tecnici in giro per il Paese. L'altra gamba della nostra lotta è ovviamente anche quella dei giornalisti coraggiosi che denunciano le malefatte che scoprono e che poi si vedono intimiditi con querele milionarie e azioni giudiziarie pretestuose o, addirittura, vengono assassinati, come successo alla giornalista Daphne Galizia a Malta due giorni fa, assassinata perché denunciava la corruzione nel suo Paese. Ma questo è il dibattito di una prossima occasione.

alla corruzione del 2014 siamo stati richiamati perché la normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione nel nostro Paese aveva un carattere generico e non sufficientemente esaustivo, non essendo in grado di coprire

In ultimo, una grave lacuna che oggi avremmo potuto colmare in modo definitivo e puntuale, ma non riusciamo a farlo, introducendo poco più che un titolo, riguarda le tutele dei segnalanti nel privato.

i ruoli di responsabilità e approfittando di benefici legati al ruolo e non certo alle persone. Personalmente ho presentato un disegno di legge in cui

e unitaria che potrebbe anche risolvere i dubbi che sicuramente si annidano nell'animo di chi - magari - ha un atteggiamento favorevole o prudenziale, come ho sentito dire dai colleghi della Lega

che potrebbe anche essere molto lungo e difficile, mentre il segnalante avrebbe bisogno di tutele nell'immediato. Anzi, oserei dire che il segnalante ha bisogno di rassicurazioni per potersi sentire tranquillo nella sua segnalazione. Spesso il segnalante si ritrova in una condizione in una condizione subalterna rispetto a soggetti che possono applicare contro di lui qualunque forma di ritorsione. Allora potremmo dire che solo i ricchi, solo chi ha una disponibilità economica si potrà permettere di segnalare? Purtroppo, se il Governo non si attiverà nella creazione di un fondo, il dubbio è reale. L'onestà sempre più spesso, nel nostro Paese, diventa monopolio di chi se la può permettere. Vogliamo dare questo messaggio? Mi rivolgo alla rappresentante del Governo.

signor relatore, l'emendamento che io avevo presentato per introdurre delle procedure chiare nel settore privato aveva ricevuto il suo parere favorevole. Chissà cosa è successo, poi, al di fuori della discussione trasparente all'interno dalla Commissione. Cosa preoccupa?

dato una dimensione plastica e tangibile di quali siano le paure. Temo che queste paure siano anche legate a una riserva nel vedere un coinvolgimento autentico e democratico della cittadinanza in un percorso di affermazione della legalità. Credo che questa sia una legge fatta prima di tutto per i giovani. I segnalanti sono soprattutto giovani, che quindi si bruciano anche la possibilità di avere davanti una carriera o un riconoscimento. Purtroppo oggi in questo Paese non succede quanto avviene negli Stati Uniti, dove i segnalanti sono considerati soggetti affidabili, a cui volentieri si affida un lavoro nelle proprie aziende. In Italia no: i segnalanti sono ancora visti con sospetto. È una legge per i cittadini, è una legge profondamente democratica, anche se incompleta. È una legge che cerca di vincere il pregiudizio negativo di chi immagina che solo nella gerarchia ci sia la salvaguardia del buon funzionamento del lavoro. Ho sentito parole che facevano riferimento al valore di una gerarchia. Bene,

possa restituire. Cosa c'è di buono? C'è di buono il fatto di avere dato sicuramente nel pubblico qualche strumento in più. C'è di buono il fatto che nel comma 5 si richiamano esplicitamente quelle linee guida dall'ANAC alle quali si spera che poi, nell'attuazione di questa legge, si possa fare pieno riferimento. C'è di buono l'inversione dell'onere della prova. Resta però molto fumoso lo scenario, perché avremo un giudice del lavoro che si troverà con la necessità di stabilire se la persona

Per questa ragione, sento di poter dichiarare il voto favorevole non solo della sottoscritta e dei tanti senatori del Gruppo Misto che non sono iscritti a componenti o che sono rappresentanti di singole componenti, ma lo dichiaro anche componenti più consistenti del Gruppo di cui faccio parte, che sono Sinistra Italiana-SEL, Italia dei Valori

Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate, innanzitutto consentitemi di approfittare di questa occasione per ringraziare tutti quei cittadini che la settimana scorsa hanno deciso di presidiare piazza Montecitorio per dire no a una legge elettorale truffa. che in un giorno feriale hanno deciso di intraprendere anche un lungo viaggio, in alcuni casi, per poter esprimere il loro dissenso e che, ancor più numerosi, la settimana prossima faranno sentire la loro voce fuori dal Senato. A loro va tutta la mia riconoscenza e a loro dovrebbe andare la riconoscenza di tutto il Paese: loro ci hanno messo la faccia. Ci hanno messo la faccia come tanti altri cittadini vorrebbero fare per denunciare la corruzione, ma oggi non hanno tutele. «Smetti di fare l'inglese, fai l'italiano». «Smetti di fare l'inglese, fai l'italiano». Signor Presidente, questa è la frase che racchiude tutto il marcio del nostro Paese. È stata la risposta che Philip, dell'Università di Firenze, si è sentito dare da uno dei suoi professori dopo aver denunciato le irregolarità. Capite bene? «Faccia l'italiano»: questa frase dovrebbe farci vergognare, eppure è la realtà del nostro Paese. Non esiste ancora una legge che tuteli chi denuncia la corruzione e il malaffare. Questa legge sarà approvata in questa sede ma dovrà passare il vaglio della Cerchiamo di capire e far capire di cosa stiamo parlando. Questa legge serve per tutelare - l'obiettivo principale è quello, non altro - chi denuncia la corruzione e il malaffare nella pubblica amministrazione. Spesso chi denuncia viene messo da parte, mobbizzato, rischia ritorsioni, viene spinto a tacere, a far finta di nulla, oppure viene additato come spia, spione, sbirro, traditore. Dobbiamo cambiare il modello culturale di questo Paese. In Italia non esiste un termine per definire chi denuncia la corruzione per porre fine al malaffare e portare onestà. Dobbiamo ricorrere a un termine inglese e anche questa è una cosa di cui dovremmo vergognarci. Li chiamiamo *whistleblower*, usando un termine inglese, perché non siamo riusciti a trovare un termine appropriato. Nel dizionario italiano non esiste una parola che possa tradurre il *whistleblowing* e dare il senso positivo di una buona pratica e questo la dice lunga sul percorso che dobbiamo ancora affrontare. Questa legge, vorrei ricordare, porta la firma del Movimento 5 Stelle: non siamo quelli del no, ma siamo anche quelli delle proposte serie e concrete. Vorrei ancora una volta rimarcare il ruolo del Senato, tanto vituperato da una parte della maggioranza che voleva abolirlo, che oggi, invece, si è trovato, fortunatamente, a

Questo Senato, a breve, si troverà a votare anche la legge elettorale truffaldina. Avevo scritto «a discutere» nel testo del mio intervento, purtroppo ho dovuto correggere «a votare» perché la discussione è stata ammazzata. Dicevo che questo Senato si troverà a votare la legge elettorale truffaldina. Dimostriamo di non essere una Camera di vassalli; riprendiamoci il ruolo che spetta a quella che è chiamata la Camera Alta e, anche per la legge elettorale, non abdichiamo al ruolo che la Costituzione ci dà. Abbiate il coraggio di fermarla e modificarla, di correggerne le storture. Tornando a noi e a questa legge, la corruzione è la peggiore piaga di questo Paese; serve il coraggio di denunciare e di metterci la faccia. Vorrei ricordare a tutti l'importanza epocale che ha avuto la legge sui testimoni di giustizia; non mi riferisco ai pentiti (quelli chiaramente hanno un altro tipo di profilo), ma a coloro che assistono o sono vittime di reati mafiosi; alle tutele riservate, ad esempio, a chi denuncia la richiesta di pizzo. Sono quelle leggi che hanno dato una svolta definitiva alla lotta antimafia. Lei, signor Presidente, dall'alto del suo ruolo di alto magistrato antimafia ricorderà sicuramente il ruolo essenziale di quelle leggi nella lotta alla mafia. mafia. Oggi la corruzione è il cancro di questo Paese, come la mafia; anzi, la mafia si nutre di corruzione e la corruzione si nutre di mafia. I due aspetti si intrecciano e anche chi denuncia fenomeni corruttivi deve avere la tutela che gli spetta. *(Applausi Questa legge potrebbe essere la chiave di volta, la svolta epocale che tutti aspettavamo. Se a questo potessimo unire l'agente provocatore, che più di una volta abbiamo provato a introdurre, creeremmo la base necessaria per estirpare definitivamente la corruzione dal Paese.

voteremo convintamente a favore di questa legge che, come dicevamo, rispetto alla versione licenziata dalla Camera ha visto corrette le storture. Oggi si presenta come una buona legge da cui partire per la tutela di chi denuncia la corruzione. Solo mettendola in atto potremo verificare le necessarie correzioni per migliorarla. Noi e tutti i cittadini onesti

per fugare ogni dubbio che questa legge sia il prezzo da pagare perché qualcuno possa votare la legge elettorale.

ringrazio tutte le associazioni e i cittadini che hanno sottoscritto le varie petizioni e che in questi anni hanno fortemente voluto e insistito per avere finalmente una legge che tutela chi denuncia il malaffare nella pubblica amministrazione. *(Applausi dal Senatore Crimi, il suo intervento mi ha dato modo di vedere accanto a lei il senatore Airola, che è stato impossibilitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea per qualche mese per una vile e grave aggressione subita e non per procedimenti che riguardano l'ordinato svolgimento dei lavori d'Assemblea. Gli diamo il bentornato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa legge che, se diverrà tale, lo sarà per il voto determinante del Gruppo del Partito Democratico lo voglio subito dire - con la consapevolezza dei suoi limiti, sul piano dell'etica amministrativa e politica non dà lezioni, ma non ne prende. Questa legge, se si esce poi dalla retorica demagogica di certe affermazioni,

fondamentale della moralizzazione della vita sociale, più che della vita pubblica. La corruzione o il malcostume, infatti, prima di avere rilievo penale, si sviluppano purtroppo nella dinamica di rapporti che sfuggono a questa dimensione e a questo rilievo. È lì che c'è la necessità di avere un meccanismo che consenta quel tipo d'informazione, che possa mettere chi ha la responsabilità della gestione di un'azienda o di un ente pubblico in condizione di fermare i fenomeni degenerativi nell'azione pubblica o in quella privata. Ben sapendo per altro che la corruzione è un fenomeno che coinvolge quasi sempre il pubblico e il privato e quindi, sotto questo profilo, la necessità è di operare tanto in un ambito, quanto nell'altro. Questo

che tale disegno di legge nasce in un quadro ordinamentale già incanalato su questa tematica, per offrire maggiori garanzie nel settore pubblico e per disciplinare nel settore privato il tema della segnalazione nell'interesse generale. Vorrei qui sottolineare che si tratta di una segnalazione, non siamo nell'ambito della *notitia criminis* data alle procure. Siamo nell'ambito di una segnalazione di un disguido e di un comportamento che può apparire anomalo e può nascondere un fatto rilevante dal punto di vista penale, ma anche delle relazioni

Sotto questo profilo, si è posto un altro tema: nel dibattito si è detto che non c'è sufficiente garanzia per il denunciato.

evidenzia le sanzioni per il denunciante che si avvalga di questa norma strumentalmente in senso negativo, costituisca una garanzia per lo stesso denunciato, che peraltro ha altri strumenti per tutelarsi, qualora la segnalazione abbia un rilievo anche di natura pubblica o venga resa pubblica. mio parere, tali considerazioni bastano a giustificare il voto favorevole del Partito Democratico, che è un voto consapevole

di essere una forza politica che lezioni di etica politica non ne prende da nessuno e non deve darle a nessuno. altrettanto consapevoli che, se questo provvedimento va al voto finale e all'approvazione, il merito è del PD e non di altri.

che segnalano tali irregolarità, dando un contributo concreto a estirpare comportamenti scorretti nell'ambito della pubblica amministrazione, vadano tutelati. Non crediamo, però, che il testo proposto raggiunga questi obiettivi, in quanto può lasciare spazio a segnalazioni di carattere strumentale che danno modo a chi le effettua

non c'è alcuna richiesta di determinatezza delle accuse e delle segnalazioni. L'indeterminatezza rischia pertanto di creare cattivo funzionamento e strumentalizzazione di ciò che viene proposto in questo testo un ulteriore rallentamento dei processi della pubblica amministrazione. Per questa ragione, esprimiamo un voto contrario al disegno di legge all'esame, proprio perché siamo favorevoli a una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. La pubblica amministrazione deve anzitutto pensare a fornire servizi in modo efficiente ed equo ai cittadini,

dichiaro la mia ferma contrarietà a questo provvedimento. Una contrarietà convinta e motivata dal fatto che esso è orientato esclusivamente alla tutela di colui che, nelle pubbliche come nelle private attività, segnala presunte patologie. Le norme non tutelano, invece, l'esigenza di stabilità delle funzioni pubbliche e delle attività produttive dalle accuse temerarie che producono effetti traumatici immediati, a fronte di una verifica circa la loro fondatezza spesso realizzata nel lungo periodo. L'assenza di un equilibrio nella disciplina può essere devastante. In particolare nelle pubbliche amministrazioni, ove è quasi sempre assente il buon datore di lavoro, possono scatenarsi sentimenti di invidia e di rivalsa con la pratica conseguenza di compromettere il bene pubblico che ne dovrebbe costituire lo scopo. Dio ci scampi e liberi dal principio innaturale *fiat iustitia et pereat mundus*. Sono infine preoccupato dal fatto che, per mere ragioni opportunistiche, molte colleghe e molti colleghi probabilmente si accingono a votare il provvedimento pur condividendo fino in fondo le considerazioni che ho qui espresso.

Le ragioni sono semplici e chiare: è un disegno di legge incostituzionale per evidenti limitazioni al diritto alla difesa che deve essere sempre garantito. Una deroga a questo diritto, garantito dalla nostra Costituzione, fa passare un ordinamento penale in uno Stato democratico a un ordinamento non democratico. Signor Presidente, coloro che dicono che chi non vuole questo provvedimento è a favore di un ammorbidimento della lotta contro la corruzione mistifica: noi siamo per una lotta senza quartiere contro la corruzione, contro il malaffare in generale, le mafie ed il terrorismo, ma riteniamo che uno Stato democratico debba farlo nel pieno rispetto dei saldi principi costituzionali che nel nostro ordinamento non possono avere cedimenti. Troppe volte si è fatta, in questi anni, deroga a questi principi di fondo, salvo poi piangere lacrime di coccodrillo dopo il sanzionamento della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Stato in cui è doveroso fare il proprio dovere - lo ribadisco - senza essere premiati, perché il proprio dovere deriva dal rispetto della legge e della sua applicazione. Allo stesso credo che non dobbiamo accettare l'idea che ci siano troppi Don Abbondio in giro, perché non ne abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno neanche di bravi, nel senso manzoniano del termine, né di innominati

Grazie